Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, in realtà la risposta all'interrogazione del senatore Vita sarà molto breve. Mi riferisco all'interrogazione n. 3-01099, presentata alla fine del 2009, con la quale si chiedono notizie in merito all'allora disegno di legge in materia di enti lirici, nell'ambito del quale egli lamenta il possibile inserimento di disposizioni sul consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia. Segnalo a tale riguardo che il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, poi convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma l, della legge 29 giugno 2010, n. 100, attualmente in vigore, non reca alcuna disposizione relativa al consiglio dì amministrazione della Biennale di Venezia.

Dicasteri competenti (o che fanno le parti di quelli competenti ) e attività ispettiva dei parlamentari. L'interrogazione 3-01099 fu pubblicata il 22 dicembre 2009, quando aveva un senso, perché era stata annunciata in modo piuttosto insistito l'ipotesi che all'interno di un decreto che doveva occuparsi di ben altra questione sarebbe stato inserito anche il punto concernente il consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia. Poi non accadde, anche perché l'opposizione fece pesare l'incongruenza e l'assurdità di un eventuale *mixage* tra temi e questioni diverse. È chiaro che l'interrogazione, con una risposta più veloce, avrebbe avuto forse un ruolo diverso, mentre ora pare una sorta di lettura *ex post*.

con riferimento all'interrogazione a prima firma del senatore Pedica, con la quale si chiedono notizie in merito al degrado di alcune vie del centro storico di Roma dovuto alla presenza di attività commerciali, sosta selvaggia e occupazione impropria di suolo pubblico, preciso che il Codice dei beni culturali e del paesaggio - cosiddetto Codice Urbani (decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42) - considera beni culturali quei beni mobili e immobili «di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico che costituiscono testimonianze aventi valore di civiltà» e beni paesaggistici gli immobili e le aree «costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio». Il patrimonio culturale della Nazione, memoria della comunità nazionale e del suo territorio, è costituito dall'insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali debbono concorrere ad assicurarne la conservazione, la pubblica fruizione e la valorizzazione. La tutela consiste nell'individuare i beni che costituiscono il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per i fini di pubblica fruizione; l'esercizio della tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, restauro manutenzione (intesa come mantenimento dell'integrità e dell'efficienza funzionale del bene). Tuttavia, per il principio di sussidiarietà verticale sancito dalla Costituzione, la disponibilità dei luoghi della cultura, nonché le attività amministrative di sorveglianza, sono svolte dall'entità territoriale

è opportuno ricordare che sia piazza Farnese che piazza Navona sono aree nelle quali è fortemente regolamentato il transito degli autoveicoli e che, a norma di regolamento del traffico cittadino, la sosta è interdetta. Il rispetto di tali prescrizioni rientra nelle competenze proprie della polizia municipale. Ad ogni buon fine si segnala che l'amministrazione comunale presenterà a breve un progetto di ulteriore limitazione al traffico, già condiviso con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio. Per quanto attiene ai lavori di restauro della fontana dei Quattro fiumi di piazza Navona, l'azione del Ministero, sempre attraverso gli uffici sul territorio, è relativa all'alta sorveglianza sulla conduzione e sulla direzione dei lavori, poiché la fontana afferisce al demanio comunale.

il senatore Augello sostiene che dovrebbero essere gli enti territoriali e, quindi, la polizia municipale a vigilare e a verificare quel degrado

sulle problematiche attinenti la gestione degli storici studi cinematografici di Cinecittà e sul supporto dei Ministero per i beni e le attività culturali alla produzione di cinema ed audiovisivo. I senatori interroganti riferiscono che, a seguito della privatizzazione, gli studi cinematografici in questione verserebbero in gravi condizioni di crisi, sia economica che occupazionale, a causa di un progressivo innalzamento dei costi e dei servizi, una sempre più accentuata esternalizzazione dei lavori, prima svolti a Cinecittà, di una sempre più ridotta competitività di mercato e della mancanza di una reale proposta per il rilancio produttivo di Cinecittà. In particolare, viene sottolineato lo scarso utilizzo dei 22 teatri di posa, la progressiva scomparsa di un cospicuo patrimonio lavorativo e professionale, nonché la chiusura di tre storici locali degli stabilimenti: la fabbrica di sculture, la tappezzeria ed il vivaio. Altre riferite Altre riferite problematiche attengono alle modalità e alle finalità del piano di sviluppo di Cinecittà Studios SpA, società che gestisce gli studi cinematografici. Posso riferire al riguardo quanto segue. Cinecittà Luce SpA (già Cinecittà Holding SpA), che ha incorporato nel maggio 2009, tramite fusione, la controllata Istituto Luce SpA, è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti patrimoniali, statutari e finanziari. Cinecittà Luce SpA è la proprietaria delle aree e degli studi cinematografici, ossia del complesso cinematografico di Cinecittà. Le attività di gestione degli studi cinematografici sono state privatizzate nel 1997 con la costituzione di Cinecittà Studios SpA. Tale società operativa ha la gestione degli studi cinematografici ed è a capitale prevalentemente privato (della Italian Entertainment Group SpA); ad essa partecipa come azionista al 20 per cento la stessa Cinecittà Luce SpA che, come già rappresentato, è l'unica proprietaria del complesso immobiliare di Cinecittà. Sin dal 1997 la gestione degli studi cinematografici è stata affidata a Cinecittà Studios SpA mediante un contratto di affitto di ramo d'azienda di Cinecittà Holding (l'attuale Cinecittà Luce); con un contratto di locazione, contestuale e separato, Cinecittà Studios SpA è locataria anche del complesso immobiliare dove sorgono gli stessi studi cinematografici. Nel 2008 la società Cinecittà Studios ha approvato un piano industriale che prevedeva, tra l'altro, un aumento di capitale in denaro da parte degli azionisti privati ed il contestuale aumento di capitale mediante conferimento del ramo d'azienda "Esercizio studi cinematografici" da parte dell'azionista pubblico Cinecittà Luce. Al perfezionamento dell'aumento di capitale, quindi, Cinecittà Studios ha acquisito tra i propri *asset* il ramo d'azienda precedentemente locato e Cinecittà Luce ha potuto incrementare la propria quota e, quindi, il valore complessivo della partecipazione, fino al 49 Successivamente, all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, Cinecittà Luce, per ottemperare al disposto della legge finanziaria 2007 in materia di partecipazioni pubbliche e tutela della concorrenza, ha progressivamente ceduto parte di questa partecipazione, attestandosi ad oggi al 20 per cento del capitale, con un accordo già sottoscritto per la completa uscita dal capitale di Cinecittà Studios entro il 2011. Sempre nel 2008, contestualmente all'aumento di capitale mediante conferimento del ramo d'azienda, Cinecittà Luce ha rinnovato il contratto di locazione immobiliare con Cinecittà Studios, prolungandone la durata, incrementandone il canone e concludendo tutte le pendenze esistenti fino a quel momento, con conseguente immediato beneficio economico e finanziario. Inoltre, Cinecittà Luce ha rinnovato il contratto, già esistente anch'esso dal 1997, di licenza del marchio Cinecittà in favore di Cinecittà Studios medesima, migliorandone le condizioni economiche e di tutela giuridica. Entrambi i contratti in questione, sono stati rivisti alla luce di esigenze di razionalizzazione economica e produttiva, con l'approvazione dei Ministeri interessati. è stato quello di porre le necessarie basi per un'articolata strategia di razionalizzazione, rilancio e snellimento delle strutture operative; il tutto per la salvaguardia e la tutela anche dei peculiari profili di interesse storico, artistico e culturale che rendono il comprensorio di Cinecittà un *unicum* al mondo.

unità produttive e centri di ricerca, rinnovando in tal modo una funzione aggregante e sistemica degli *studios*, in ogni sinergia possibile con le imprese del settore. Tale Distretto potrà ospitare circa 150-200 tra piccole e medie imprese, studi professionali, centri di formazione e ricerca. È del tutto evidente, quindi, come questo progetto vada a rafforzare e valorizzare tutta la struttura degli studi cinematografici, oltre a porre le basi di concrete prospettive occupazionali, e costituisca un investimento nei settori tipici e peculiari del comprensorio dì Cinecittà, con l'aggiunta di indispensabili servizi di supporto. In merito alla riferita chiusura di tre storici locali di Cinecittà, si fa presente che tale misura ne riguarda due - la fabbrica di sculture e stucchi della società Cinears e la tappezzeria della società Sanchini ed è la conseguenza di recessi contrattuali operati da Cinecittà Studios, che ha in locazione gli studi cinematografici ed è titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i contratti con le società Cinears e Sanchini. Tali scelte, che esulano dalla sfera di competenza di Cinecittà Luce SpA, si collocano nell'ambito delle ordinarie attività svolte da un'impresa commerciale. Cinecittà Studios ha peraltro, su richiesta di Cinecittà Luce, fornito elementi in merito ai motivi che hanno determinato tali scelte imprenditoriali, imprenditoriali, rappresentando che le disdette operate sono ascrivibili essenzialmente a morosità protratte nel tempo e che, in particolare per la società Cinears, i rilevanti spazi occupati (5.000 metri quadri, di cui circa 2.000 metri quadri coperti) si trovano in situazione di degrado quanto a conservazione dei materiali e sicurezza dei capannoni. Inoltre, le attività sia della Cinears che della Sanchini hanno subito, nel corso degli anni, un drastico ridimensionamento ed un mancato adeguamento alle moderne esigenze del mercato. Le disdette sono state comunicate con un anno di anticipo e pertanto avranno effetto solo nel maggio 2011; si precisa che nessuna disdetta contrattuale ha interessato il vivaio. Sottolineo, da ultimo, come lo stanziamento per il Fondo unico per lo spettacolo risulta determinato, per il triennio corrente, dalla tabella C della legge di stabilità per il 2011, in misura notevolmente ridotta rispetto a quella autorizzata per il 2009, risultando pari a 258,6 milioni di euro. Nel 2010 i fondi stanziati per il funzionamento di Cinecittà Luce sono stati pari a 17 milioni di euro, di cui 12,2 milioni derivanti dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e 4,8 milioni derivanti dai fondi del Lotto. Cinecittà Studios SpA dal 1997, anno della privatizzazione, ha ospitato la realizzazione di ben 27 produzioni internazionali (ricordiamo, tra le altre, «Gangs of New York» di Martin Scorsese, «La passione di Cristo» di Mel Gibson, la serie tv «Roma», prodotta da HBO, «Miracolo a Sant'Anna» di Spike Lee) e di oltre 40 film italiani; nei suoi teatri di posa sono state inoltre girate 40 serie annuali delle principali *fiction* televisive italiane. Attraverso una politica di acquisizioni e di crescita, oggi Cinecittà Studios SpA assomma 4 centri di produzione (2 a Roma, 1 in Umbria e 1 in Marocco) e tutti i servizi di postproduzione attraverso la controllata Cinecittà Digital Factory. Nel decennio successivo alla privatizzazione, il fatturato ha visto un sostanziale raddoppio rispetto alla media degli ultimi anni anni ante-privatizzazione, passando da 18-20 milioni di euro a circa 40 milioni di euro. In riferimento alla competitività, si segnala che, diversamente da quanto rappresentato, essa risulta migliorata, dato che i prezzi delle lavorazioni effettuate da Cinecittà Studios sono sensibilmente diminuiti rispetto al passato attualmente (dato dell'11 ottobre 2010) i teatri impegnati sono 19. Per quanto concerne il dato occupazionale, esso è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al passato, con circa 224 occupati assunti a tempo indeterminato ed è rilevante notare che oltre la metà degli attuali occupati, ossia 120 su 224, sia stata assunta stabilmente proprio in questi ultimi anni. Tale patrimonio professionale e lavorativo è stato mantenuto nella sua varietà sia con riguardo ai profili professionali di stampo più tradizionale, quali ad esempio addetti alle scenografie e falegnami, decoratori, sia con riguardo alle nuove professionalità emergenti nel campo architettonico-ingegneristico, nell'area della postproduzione digitale e nel marketing-commerciale. Peraltro, si rappresenta che le risorse sinora investite nel complesso di Cinecittà da Cinecittà Studios sono oltre 30 milioni di euro. Ai positivi risultati sinora ottenuti si aggiunge un ulteriore traguardo, successivo al risanamento ed alla razionalizzazione e mirato allo sviluppo ed alla valorizzazione del comprensorio di Cinecittà, al fine di renderlo competitivo con le esigenze del mercato cinematografico e audiovisivo anche internazionale. Si tratta dell'accordo stipulato tra Cinecittà Luce SpA e Cinecittà Studios SpA concernente lo sviluppo immobiliare interno del comprensorio di Cinecittà. Tale accordo è stato oggetto di lunga, accurata e complessa istruttoria. Stipulato preliminarmente nel maggio 2009, e ratificato il 10 luglio 2009 da Cinecittà Luce SpA, come previsto nello stesso accordo preliminare, è divenuto efficace dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del Ministro per i beni e le attività culturali in data 4 agosto 2009, sulla base del motivato parere istruttorio reso dalla competente Direzione generale per il cinema. L'accordo in questione che, si ribadisce, ha ricevuto l'assenso del Ministero, azionista unico di Cinecittà Luce SpA, in estrema sintesi si concretizza, per la prima fase dell'operazione di sviluppo, nella cessione da parte di Cinecittà Luce a Cinecittà Studios dei diritti edificatori e nella contestuale cessione dei diritti di superficie per 39 anni a fronte di un canone determinato sulla percentuale del 15 per cento del valore complessivo dell'investimento effettuato da Cinecittà Studios. L'esigenza perseguita attiene alla valorizzazione all'interno del comprensorio dei diritti di cubatura ed al rispetto dell'ulteriore esigenza di valorizzazione prevalentemente in settori legati all'attività cinematografica tipici di Cinecittà Luce SpA. Atteso che Cinecittà Studios SpA è partecipata al 20 per cento da Cinecittà Luce SpA e che ha in essere, sempre con Cinecittà Luce SpA, un rapporto di locazione del complesso immobiliare di Cinecittà (in corso dal 1997 con scadenza nel 2026) è evidente come il suo ruolo per tale finalità di valorizzazione sia imprescindibile. La rilevante opportunità a beneficio di Cinecittà Luce SpA è ancor più evidente se si considerano due aspetti. Da un lato, il beneficio derivante dalla valorizzazione di un potenziale edificatorio fino ad oggi economicamente inespresso, senza alcun impegno di carattere finanziario da parte della società e con il successivo rientro nella disponibilità dell'intero patrimonio immobiliare al termine del periodo di concessione. Dall'altro, l'intervento di valorizzazione da parte di Cinecittà Studios prevede la realizzazione, a totale beneficio degli studi (e quindi del comprensorio di proprietà di Cinecittà Luce), di alcuni volumi edificabili, funzionali all'attività cinematografica, in spazi attualmente inutilizzati. Gli spazi e gli edifici per il settore cinematografico che si andranno a costruire resteranno quindi, dopo la conclusione del rapporto contrattuale relativo alla cessione dei diritti di superficie (39 anni), di proprietà di Cinecittà Luce SpA (e quindi dello Stato), saranno realizzati con risorse private; si precisa, inoltre, che nessun edificio storico di Cinecittà sarà interessato da queste nuove costruzioni. Pertanto, al vantaggio immediato del canone pattuito per la cessione dei diritti di superficie si aggiungerà anche l'accrescimento di valore dell'area a seguito delle edificazioni. Si evidenzia peraltro che i diritti edificatori derivano da una convenzione stipulata nel dicembre 1983 tra il Comune di Roma e l'allora Cinecittà SpA e che, dopo quasi 30 anni, presentano ora una possibilità di utilizzo economico. Tale piano di sviluppo porterà ad un incremento delle strutture necessarie alle principali attività degli *studios*: un nuovo grande teatro di posa, attrezzato con le migliori tecnologie oggi disponibili, per renderlo flessibile e modulare, adatto alle riprese cinematografiche con integrazioni digitali e 3D, nonché moderni uffici e attrezzerie necessari al funzionamento non solo al nuovo teatro di posa, ma anche di tutti gli altri teatri limitrofi. Inoltre, il piano di valorizzazione presentato da Cinecittà Studios Spa prevede la creazione

milioni derivanti dai fondi del Lotto. Simulando la ripartizione dello stanziamento del 2011 rispetto alle percentuali stabilite nel 2010, le risorse disponibili per Cinecittà Luce SpA si sarebbero assestate, verosimilmente, intorno ai 7,5 milioni di euro. Debbo tuttavia con soddisfazione comunicare che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 marzo, ha tra l'altro autorizzato un reintegro del predetto Fondo con una dotazione ulteriore di 149 milioni di euro. Con tale nuova disponibilità, assicuro gli onorevoli interroganti che saranno tenute in debita valutazione le esigenze della Società Cinecittà Luce SpA con una integrazione di fondi che consentirà lo svolgimento delle attività in base all'atto di indirizzo disposto dal Ministro in ordine alle competenze di tale struttura.

si considerano anche le sue varie e più complesse articolazioni avvenute nel corso del tempo (poi si potrà giudicare se la scelta del 1997 fu più o meno fausta quanto all'articolazione nella *holding*, con Cinecittà Studios, e così via), è quello che nel mondo, insieme all'opera lirica e ad alcune grandi produzioni culturali, fa dell'Italia - *malgré tout*, si direbbe - un Paese di straordinario peso nel villaggio globale. Basta pronunciare

che è sotteso alle nostre interrogazioni, ne è un po' il sotto testo (piano che peraltro non è noto: anzi, si tratta dell'unico punto su cui la ringrazierò in questa mia risposta, perché per la prima volta è pubblica una discussione sull'argomento, ci risulta che nemmeno le organizzazioni sindacali abbiano avuto l'opportunità di conoscere non solo e non tanto che ne sarà del lavoro - già sarebbe molto - ma anche che ne sarà della struttura dentro la quale operano)

un fatto già successo, non è la prima volta che accade. I grandi studi del cinema di Mosca hanno fatto con Putin la stessa fine, e cioè da grandi luoghi del cinema sono diventati luoghi di alberghi di lusso.

o alla famiglia De Angelis che fa anche sculture e le strutture per i tanti film che abbiamo visto, per motivi puramente di affetto, tal modo è il cinema italiano che viene distrutto. Lei sa che per ricostituire questi artigianati complessi e culturalmente così sofisticati servono molte generazioni. Ecco, siamo profondamente delusi, ma soprattutto siamo inquieti.

del sottosegretario Augello, per la risposta molto articolata, che tuttavia - mi dispiace - non è soddisfacente dal nostro punto di vista. Già il senatore Vita ha articolato le varie questioni.

dietro ad un marchio storico unico nel mondo come quello di Cinecittà - lo ripeto, unico nel mondo ripeto, unico nel mondo - non si nascondesse - lo dico brutalmente - l'ennesima speculazione edilizia mascherata per dare la possibilità ad alcuni imprenditori

sita nella X circoscrizione, che conosco benissimo avendo la fortuna di abitare proprio alle spalle

lo Stato si ritira e i privati possono speculare per il loro tornaconto, e dunque non certo per difendere la cultura o l'immagine del Paese, ma semplicemente, a mio modesto parere,

in relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dai senatori Perduca e Poretti, concernente il pagamento da parte dell'Italia delle spese per l'acqua utilizzata dalla Città del Vaticano, in conformità a quanto comunicato dall'Ufficio studi e rapporti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, faccio presente quanto segue. La questione concernente il regime idrico dello Stato Città del Vaticano è stata esaminata da un'apposita Commissione bilaterale istituita nel 2001, che ha approfondito tutti gli aspetti connessi con tale regime sulla base della lettera e dello spirito del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, in particolare dell'articolo 6, e della Convenzione attuativa del 1931. A conclusione di tali approfondimenti, la questione è stata definitivamente risolta nel 2004 e con completa soddisfazione reciproca, attraverso lo scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Cardinale Segretario di Stato, costituente un'Intesa chiarificatrice dell'interpretazione e dell'attuazione dell'articolo 6 del Trattato Lateranense. Tale articolo, infatti, prevede che sia assicurata alla Città del Vaticano una adeguata dotazione di acque in proprietà e che sia altresì assicurato il coordinamento dei servizi pubblici alla stessa connessi. Nell'Intesa si riafferma il principio della gratuità della fornitura di acqua alla Città del Vaticano, sia all'interno delle Mura Leonine che all'esterno, a beneficio delle sedi di Dicasteri e degli enti centrali della Chiesa indicati dalla Santa Sede in un apposito elenco. La Santa Sede continua, comunque, a corrispondere all'ACEA un contributo periodico in riconoscimento degli oneri connessi con il trasporto dell'acqua, già erogato sulla base della Convenzione del 1931 e della Convenzione del 1982, attuata da una prassi consolidata e parte integrante della nuova Intesa. In base ad essa, inoltre, la Santa Sede ha versato all'ACEA, a titolo di contributo *una tantum* per i costi di gestione delle risorse idriche che gravano sull'ente erogatore, una somma corrispondente al costo della costruzione di un depuratore, pari a 1.100.000 euro. Nella legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003 n. 350) è stata introdotta una norma volta a porre fine alla controversia con l'ACEA, in base alla quale il Ministero delle infrastrutture ha erogato una somma pari a circa 20 milioni di euro, corrispondente al debito vantato dalla società erogatrice per il passato, e versa dal 2005 una somma annuale non superiore a 4 milioni di euro per i costi di depurazione delle acque. del 23 aprile 2004, emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Modalità, criteri ed ammontare del contributo compensativo a carico del bilancio dello Stato, da corrispondere ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei soggetti creditori per la fornitura dei «servizi idrici» dello Stato Città del Vaticano» sono state disciplinate le modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni.

ciò che sarebbe al centro della interpretazione a seguito dei lavori della famosa Commissione. Infatti, se è vero che l'Italia deve provvedere, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata una adeguata quantità di acqua in proprietà, non sono state date risposte soddisfacenti relativamente allo smaltimento dei reflui, che invece ha un certo impatto dal punto di vista dell'impegno economico che si ha nei confronti dello dello Stato Città del Vaticano in virtù del Concordato. Avevamo anche chiesto di capire se e come - essendo tra l'altro in questi mesi aperto in Italia un dibattito relativamente all'acqua per quanto attiene sia alla proprietà che al bene pubblico che essa rappresenta - vi siano in corso campagne relative al contenimento del consumo idrico. Negli ultimi mesi si sono anche verificati fatti che vanno al di fuori della legge e che credo debbano essere presi in considerazione. Sappiamo che, senza alcuna autorizzazione, il Vaticano sta costruendo un palazzo accanto a San Paolo, con tanto di *auditorium*, e sta ingrandendo i padiglioni dell'ospedale «Bambino Gesù». Siccome ci si avvale dell'immunità diplomatica, i vigili urbani non possono entrare nei cantieri per verificare cosa stia succedendo. Tutto ciò è contro la legge, perché sono veri e propri abusi edilizi. Noi, come Stato italiano, continueremo a pagare attraverso questa bolletta (che, come mi pare di capire, non viene non viene calcolata necessariamente sulla quantità di acqua consumata, ma sulla base di indennizzi forfetari nei confronti dell'ACEA) anche la fornitura di acqua in questi luoghi,

non si volessero aggiungere quelli che dal 2005 sono stati forniti ad integrazione. Ripeto però che resta il problema di arrivare a un'interpretazione - non so se dovremo presentare un'altra interrogazione parlamentare al riguardo - per capire il perché si ritenga che nell'acqua in proprietà debbano rientrare anche i reflui: francamente si stenta a capire quale possa essere il nesso di questo tipo di interpretazione, a meno che non si voglia continuare a far pervenire determinati finanziamenti

e nello stesso tempo di un'occasione per perseguire la necessità di rendere quanto più trasparenti i nostri rapporti interni, e anche quelli esterni con i fornitori, mi rimetto ancora una volta alla sua benevolenza per avere un'informazione al riguardo. L'anno scorso il bilancio preventivo del Senato è stato discusso a metà settembre: ciò non dovrebbe avvenire mai, e sicuramente non a seguito di una serie ripetuta di richieste di informazione circa la data della consegna di tale documento.

Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze*: «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo»